con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato per la salute il sig. Luca COLETTO.

mercoledì 5 dicembre, sono nuovamente convocate, per la loro costituzione, mercoledì 12 dicembre, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario, secondo gli orari di seguito indicati: - ore 8,30: Commissione parlamentare per la semplificazione e Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria; - ore 14: Commissione parlamentare per le questioni regionali e Commissione parlamentare di controllo

del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti VIII, nn. 1 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017) 2017) e 2 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018). Il relatore, senatore Pesco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

Signor Presidente, alla riunione dei Presidenti di Commissione (che, in base al Regolamento, presiedo in quanto Presidente della Commissione bilancio) il Collegio dei Questori ha presentato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017 e il progetto di bilancio preventivo per l'anno finanziario 2018. Vorrei riportare i dati essenziali di questi documenti contabili, mentre saranno i senatori Questori a illustrarli nel dettaglio. Iniziamo da un raffronto tra la spesa a consuntivo del Senato nel 2012 e quella nel 2017. Nel 2012 essa era pari a circa 520 milioni di euro al netto dei risparmi, mentre nel 2017, sempre al netto dei risparmi, risulta pari a circa 488 milioni di euro. Vi è stata, dunque, una riduzione, nell'arco di pochi anni, di oltre

Si tratta senz'altro di un risultato notevole per l'Amministrazione del Senato, tenendo conto che questa contrazione della spesa non ha determinato uno scadimento nella quantità e qualità dei servizi offerti, all'innovazione tecnologica e organizzativa e, dall'altro, all'impegno profuso dall'Amministrazione, nonostante la consistente riduzione del personale in servizio registrata nell'arco temporale indicato. Questo è un risultato che può quindi riempire di legittimo orgoglio la Presidenza del Senato, i senatori Questori, il Segretario Generale e tutta la macchina del Senato. Il Senato ha dunque fatto la sua parte, negli anni passati, all'interno del processo di risanamento della finanza pubblica. È legittimo affermare che la seconda istituzione della Repubblica ha partecipato in maniera significativa al percorso di contenimento della spesa che ha interessato anche le altre amministrazioni dello Stato e possiamo promettere che la nuova politica economica che sarà portata avanti dall'attuale maggioranza politica non devierà, relativamente alla spesa di Palazzo Madama, dal percorso di parsimonia e - soprattutto - efficienza finora compiuto. Per quanto riguarda la composizione della spesa, quella di funzionamento è risultata pari, nel 2017, al 54,37 per cento della spesa complessiva, contro il 45,63 per cento della spesa previdenziale, intesa come somma della spesa previdenziale per gli *ex* senatori e di quella per egli ex dipendenti del Senato, che notoriamente è ricompresa nel bilancio di ciascuna delle due Camere.

Per il resto, la tabella n. 5 del rendiconto 2017 (Quadro riepilogativo finale della spesa obbligatoria), che ci mostra il costo dell'attività politica vera e propria del Senato (ovvero quello dei senatori e dei Gruppi parlamentari), ci informa che tale spesa risulta nel 2017 in diminuzione rispetto al 2016. È questa, peraltro, una spesa di cui si poteva apprezzare la riduzione, sia pure contenuta già nel rendiconto 2016, in rapporto al rendiconto 2015. Per quanto riguarda il trattamento del personale dipendente di ruolo, nel rendiconto 2017 si registra una riduzione della spesa rispetto all'anno precedente, dove essa risultava a sua volta in calo rispetto al 2015. Peraltro, tale voce di spesa risulta in diminuzione anche nel bilancio di previsione 2018 rispetto all'esercizio 2017. Al riguardo, occorre evidenziare che la riduzione della spesa relativa al personale dipendente di ruolo rappresenta, almeno in parte, l'effetto contabile della riduzione del numero dei dipendenti in servizio, in corso ormai da diversi anni. Le misure adottate per l'anno 2018 hanno in parte frenato questa emorragia, così come, sotto altro profilo, ha frenato la tendenza alla riduzione della spesa in parola; ma è chiaro che, in prospettiva, dobbiamo interrogarci sull'esigenza di dare avvio a nuove procedure di concorso, al fine di stabilizzare quantomeno il numero dei dipendenti del Senato su una cifra compatibile con il buon andamento dell'amministrazione. Naturalmente la questione del personale può anche essere esaminata nel quadro di una razionalizzazione degli Uffici. L'esigenza di prevedere, in futuro, un aumento della spesa in relazione allo sblocco del *turnover*, con le relative nuove assunzioni, potrà infatti essere affrontata anche in un'ottica di semplificazione complessiva, tenendo conto delle sinergie conseguibili grazie alla realizzazione dei poli parlamentari. Su questa strada, che già ha consentito di realizzare importanti risparmi negli anni scorsi, credo si dovrà proseguire anche in futuro, in modo da razionalizzare il funzionamento della macchina amministrativa delle due Camere. Ricordo inoltre che al bilancio delle Camere affluisce anche il finanziamento statale destinato all'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito a seguito della riforma dell'articolo 81 della Costituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Tale norma prevede infatti uno stanziamento 3 milioni di euro, che lo Stato versa a ciascuna Camera, affinché venga destinata alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio. Questo è il quadro generale del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2017 e del progetto di bilancio preventivo per l'anno finanziario 2018. Quest'anno, come già avvenuto cinque anni or sono, il cambio di legislatura non ha consentito di esaminare i predetti documenti contabili prima della pausa estiva. Come è noto, tuttavia, il ritardo ha consentito di apportare, a parità di spesa complessiva, alcune limitate modifiche al bilancio di previsione per l'anno in corso, che era stato precedentemente deliberato dal Consiglio di Presidenza sul finire della scorsa legislatura. Le modifiche riguardano da un lato l'aumento degli stanziamenti per alcuni articoli, nella prospettiva di rafforzare le attività interparlamentari e internazionali del Senato e quelle di ricerca e di documentazione, nonché di valorizzare e sviluppare ulteriormente l'aggiornamento professionale del personale e le politiche di pari opportunità; dall'altro, l'istituzione di nuovi articoli, con i relativi stanziamenti, al fine di promuovere investimenti relativi ai Palazzi, volti al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione, efficientamento energetico e tutela ambientale, eliminazione delle barriere architettoniche e riqualificazione delle aree esterne adiacenti agli stessi.

Presidente, colleghi, grazie per

piacere, perché significa che l'attenzione che abbiamo voluto dare al funzionamento del Senato in tutti i suoi aspetti, sia da un punto di vista legislativo, relativo ai lavori dell'Aula, sia da un punto di vista amministrativo, per quanto riguarda la conduzione della vita all'interno del nostro contesto quotidiano, ha rappresentato un fattore positivo. Il bilancio di previsione per il 2018 era stato approvato già nello scorso 14 marzo,

chiaramente in accordo con l'amministrazione comunale romana, di riqualificazione delle aree adiacenti ai nostri Palazzi, in maniera tale da

La trasmissione telematica degli atti parlamentari mediante firma digitale è un altro progetto in cantiere per un Senato con sempre minori sprechi cartacei. Il processo di dematerializzazione è già in atto con il 75 per cento di carta in meno e con 4,6 milioni di euro risparmiati.

degli ordini del giorno in merito, ma proprio per questo nostro impegno non sono stati presentati. Ringrazio i presentatori che ci hanno dato fiducia in questo percorso. Passo all'illustrazione dei documenti contabili oggi all'esame e agli aspetti burocratici e amministrativi, ma importanti del rendiconto delle entrate e delle spese per l'anno La spesa complessiva del Senato, al netto dei risparmi riversati, ammonta a 488.930.460,71 euro,

le somme versate direttamente dai senatori c'è una conduzione attenta e precisa, mese per mese, proprio per tranquillizzare sul fatto che la gestione delle risorse pubbliche e private è perfettamente in regola e trasparente rispetto a quanto ci viene chiesto. Se guardiamo alla spesa del Senato, possiamo notare che le spese di funzionamento generale occupano il 55 per cento del totale della spesa del Senato, con una diminuzione di 5 milioni rispetto al 2017, nonostante il cambio di legislatura. l'attenzione su questo, che è un altro aspetto importante che voglio ribadire.

al bilancio di previsione per il 2018, la spesa scende ancora a 539 milioni, quindi un altro anno in diminuzione, come ho accennato

per l'ottavo anno consecutivo registra il segno meno nelle previsioni di spesa. Nel 2018 al momento si registrano 12 milioni di euro di risparmi.

Peraltro, oltre alla minore dotazione, il Senato ha risparmiato ulteriori risorse dal 2013 ad oggi, per un totale di circa 92 milioni di euro e questo è un dato veramente importante.

I principali scostamenti di spesa rispetto alle previsioni del 2017 sono dovuti a nuove valutazioni di politiche di bilancio, ai rimborsi di natura indennitaria sostenuti per lo svolgimento del mandato parlamentare, ai servizi informatici e di riproduzione, ai trasferimenti ai Gruppi

agli ex senatori, d'altronde dal 2012 abbiamo un calcolo basato sul sistema contributivo e non retributivo, quindi si è passati a un calcolo completamente diverso. Il contributo di solidarietà,

il rinnovo delle infrastrutture informatiche sia stata compiuta una vera e propria rivoluzione digitale, grazie alla quale abbiamo realizzato un risparmio di 2,5 milioni di euro, che ha portato il Senato della Repubblica italiana a diventare

L'attività legislativa è diventata sempre più 4.0: basta pensare alla app Tabulas, alla app per le agenzie di stampa, per la rassegna stampa, per il *restyling* del sito del Senato, anche per quanto riguarda un Senato sempre più leggero, più digitale e meno cartaceo. Il contratto di riproduzione digitale ha ridotto, come dicevo, le copie

come dicevo prima, e delle Aule delle Commissioni, grazie anche al sito Open data del Senato stesso e l'implementazione della *web* TV del Senato fino a otto canali. Ad oggi, più di tre milioni di persone hanno seguito i lavori del Senato e credo che questo sia un aspetto veramente importante. importante. Il Senato è sempre più aperto anche al contributo dei cittadini al processo legislativo: lo è grazie al lavoro dell'Ufficio valutazione e impatto delle politiche pubbliche, che, tra noi

realizzato sui temi di economia e finanza. Abbiamo investito su qualità e innovazione per costruire il futuro. Più che mai oggi questo è uno degli aspetti importanti, anche per dare la possibilità di integrare le richieste,

giusto, forse era in eccesso: ma oggi è poco, e credo che questo sia uno degli aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. Le integrazioni funzionali che stiamo facendo tra Camera e Senato riguardano i poli parlamentari, i servizi sanitari, i servizi informatici e della documentazione, con l'implementazione del polo bibliotecario già esistente e degli archivi storici. A proposito di archivi storici, entro la fine dell'anno i due archivi di Camera e Senato opereranno con la stessa infrastruttura. È previsto anche uno schema procedurale, che con il senatore Arrigoni abbiamo esaminato, di gare comuni da bandire tra Camera e Senato. Parlo della gestione dei servizi informatici, dell'assistenza all'utenza, della prestampa, della rassegna stampa e del canale satellitare. Quindi, credo più che mai che questo sia il nostro punto di forza. Palazzo Madama in questi anni (e io da Questore, con i colleghi, me ne sono reso conto) più che mai è fatto soprattutto, come qualsiasi istituzione, di persone. Consentitemi, dunque, un ringraziamento di cuore a tutti coloro che con passione, professionalità e grande senso delle istituzioni lavorano in questa struttura, dimostrando all'esterno che la qualità esiste; esiste nella competenza, nella professionalità e nella motivazione dei singoli. Questo significa anche fare squadra. Credo che affinché una istituzione possa andar bene, chiaramente al di là delle valutazioni politiche differenti com'è giusto nella discussione democratica, si debba fare squadra quando ve ne è la necessità.

ci dà una mano per raggiungere questi obiettivi, perché senza di loro non potremmo farcela. Parlo in modo particolare del Segretario Generale e dei Vice Segretari Generali,

altrettanto particolare va ai nostri assistenti qui in Aula, ma non solo qui in Aula, perché ci danno una mano quando qualcuno di noi si agita un po'

bilancio previsionale che sono stati espressi in modo molto chiaro sia dal Presidente della Commissione bilancio che dal Presidente del Collegio dei Questori.

circa 222 milioni di risparmio del Senato dal 2013 al 2018.

in quell'epoca abbiamo disdetto gli uffici dell'ex Hotel Bologna, che ospitavano dei senatori, con il risparmio che si è generato successivamente. Già in quegli anni infatti abbiamo indicato la linea del blocco del *turnover*,

Forse un po' pochini; bisognerebbe rivalutare se le risorse umane siano sufficienti, posto che la riduzione del personale si poneva anche, negli ultimi anni, alla vigilia di un'ipotetica un'ipotetica cancellazione, come qualcuno la definiva, o comunque sostituzione del Senato, che sarebbe stato chiamato a svolgere ruoli più ridotti rispetto a quelli previsti dall'attuale Costituzione che - per fortuna - è rimasta immutata. Le indennità dei senatori sono scese; prima incidevano del 19 per cento sulla spesa totale del Senato, ora sono scese al 10 Le spese previdenziali sono scese di 8 milioni rispetto al 2017 e le spese di funzionamento di ben 7 milioni rispetto al 2017. Il *trend* è quindi in crescita nel senso della

dipendenti. Cosa dire del sistema della comunicazione? Nel 2017, tre milioni di italiani hanno avuto la possibilità di seguire i nostri lavori e di accedere ai siti *online*. Cosa dire della campagna della politica *green* e del contrasto a tutto quello che può essere inquinante? Pensiamo, ad esempio, alle autovetture del Senato che si autoricaricano e non vanno a gasolio o benzina.

Io sono fiero di questa Amministrazione, dei giovani che ho lasciato quando ero Presidente del Senato, e che ho trovato adesso funzionari e dirigenti, che ci vengono invidiati

un eccellente, validissimo funzionario di un'importantissima Commissione è stato chiamato a far parte di una struttura strategica dell'attuale Presidente del Consiglio - a conferma, senatori Questori, colleghi, che l'Amministrazione esprime professionalità che si pongono e sono neutre nei confronti della politica, perché vengono chiamate a dare una mano alle istituzioni, e quindi ai Governi che si susseguono, al di là

responsabile, per obbligazione di risultato, nei confronti del Presidente del Senato. Ma io penso che il risultato della nostra Amministrazione, dall'assistente parlamentare fino agli alti gradi, ci possa lasciare sereni ed entusiasti di quello che danno quotidianamente i nostri giovani e i meno giovani.

che hanno reso possibile tutto ciò. Ma ciò che, per quanto mi riguarda, è da mettere assolutamente in evidenza è

i cittadini, perché siamo il luogo per eccellenza di produzione legislativa, a questo ha un riverbero immediato e diretto. Ciò

quindi, ringrazio non solo i Questori e tutto il Consiglio di Presidenza, ma anche il Segretario Generale, la struttura del Segretariato e tutti i Direttori dei

per il lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, da parte sia della struttura politica, e quindi di tutto il Consiglio di Presidenza, che di tutta la struttura amministrativa. Chiudo con un aneddoto: quando sono entrata la prima volta in

con la propria professionalità è la vera garanzia dell'autonomia, dell'indipendenza e della terzietà, fondamentale per il nostro lavoro.

senatrici e senatori, il dibattito odierno sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato relative all'anno 2017 e sul progetto di bilancio interno per l'anno 2018 si è sviluppato in modo apprezzabile e con un confronto serio fra le diverse parti politiche di maggioranza e opposizione. Il dibattito, infatti, ha toccato molti punti inerenti alle voci di entrata e di spesa del Senato, che hanno testimoniato l'interesse e l'impegno politico dei vari Gruppi politici di maggioranza e di opposizione, affinché questa Istituzione prosegua nel percorso virtuoso intrapreso ormai da tempo e che tutti - seppure ciascuno con il proprio stile - dovrebbero perseguire e migliorare ulteriormente. Il giudizio positivo che intendiamo esprimere sul rendiconto 2017 si fonda non soltanto sui dati che emergono dal documento al nostro esame, ma anche sulle modalità con cui questi sono stati conseguiti. conseguiti. In un momento in cui sono stati chiesti sacrifici al Paese per portare sotto controllo i conti pubblici, il Senato ha notevolmente ridotto il proprio peso sulle finanze pubbliche. Nella scorsa legislatura, il Senato si è impegnato con costanza su un percorso di riduzione dei propri costi e ha migliorato i propri servizi, e il fatto che abbia mantenuto questi impegni credo sia da rimarcare con grande soddisfazione. Noi tutti, insieme a tutta la struttura del Senato, siamo stati attori e protagonisti di questo percorso virtuoso, nato con l'ormai noto ordine del giorno G100 - proposto dal PD e approvato nel 2012 che dettava per il Senato un traguardo che allora poteva sembrare ambizioso: un cambiamento di abitudini, spese e assetti organizzativi che sembravano difficili da raggiungere e che invece, con tenacia e costanza, sono stati perseguiti anno dopo anno. la macchina organizzativa dell'Istituzione è oggettivamente migliorata: i servizi, in particolare quelli gestiti insieme alla Camera, sono più efficienti ed è stata aperta la strada per nuovi e ulteriori miglioramenti. Sicuramente - come hanno già ricordato in molti - una parte consistente di questo miglioramento dell'Istituzione va riconosciuto come merito al personale dipendente, a cui sono stati chiesti i maggiori sacrifici in termini di riduzione del peso all'interno del bilancio del Senato, senza che venisse meno la qualità del servizio. Tutti insieme abbiamo sottolineato come ciò significhi una sola cosa: sola cosa: alta professionalità. Ciò che maggiormente colpisce in senso positivo dall'esame dei dati del rendiconto 2017 è che, dal 2012 al 2017, la spesa si è ridotta, al netto dei risparmi da versare allo Stato: da 520 milioni di a 488 milioni di euro circa. Fatto salvo l'incremento della spesa per il personale in quiescenza, il rendiconto 2017 presenta una riduzione in tutti i macroaggregati della spesa corrente obbligatoria (senatori e Gruppi parlamentari, ex senatori, segreterie istituzionali, personale dipendente in servizio e oneri previdenziali e fiscali) rispetto sia al 2016 sia al 2015. L'avanzo di esercizio segna un nuovo andamento positivo passando da 44,2 milioni di euro del 2015 a 59,9 milioni di euro nel 2016 e a ben 64,3 milioni di euro nel 2017. Questi pochi numeri sono importanti prima di tutto per il loro valore simbolico, ma anche per il loro numero assoluto, e assumono ancor più valore se si tiene conto del buon livello di efficienza ed efficacia raggiunto dall'Istituzione. Dato atto dei risultati positivi raggiunti, ci troviamo oggi di fronte a nuove sfide. Potremmo ritenerci soddisfatti, ma proprio da questi risultati penso dobbiamo ripartire per impostare nuovi traguardi e lasciare alla prossima legislatura un Senato ancora più efficiente. La XVIII legislatura è agli inizi e occorre Il progetto di bilancio per l'anno 2018 non contiene particolari indicazioni in tal senso, anche in ragione del passaggio tra la vecchia e la nuova legislatura. Riteniamo, tuttavia, che uno degli ambiti su cui dovremmo confrontarci nei prossimi mesi e su cui lavorare da qui alla fine della XVIII legislatura sia quello dell'intensificazione delle sinergie con la Camera dei deputati, con l'obiettivo di accentuare, quanto più possibile, l'erogazione in comune di servizi di natura identica, che ancora oggi le due istituzioni erogano ai parlamentari in modo separato. Sul tema dell'unificazione dei servizi di Camera e Senato molto ancora può essere fatto. Penso - ad esempio - al Servizio studi, che già oggi produce documenti in comune ma operando da sedi separate. Penso, poi - per fare qualche esempio - che sarebbe utile unificare i servizi informatici, quelli tecnici e di ragioneria, di rassegna stampa, i rapporti internazionali e quant'altro rimasto ancora a gestione separata. Soprattutto riteniamo indispensabile, anche per ragioni di trasparenza delle istituzioni, che sia creata una centrale unica per le gare d'appalto e i contratti. Si potrebbe lavorare, poi, per mettere insieme e gestire in comune, oltre ai servizi, anche gli immobili a disposizione delle due istituzioni, per meglio corrispondere alle esigenze del mandato parlamentare, per migliorare la qualità delle prestazioni offerte e agevolare il lavoro svolto dalle alte professionalità presenti nell'istituzione: in poche parole, condivisione delle strutture, meno Uffici e più servizi. Per quanto riguarda il personale, occorre intervenire per migliorare tutte le dotazioni strumentali necessarie ad accrescere l'efficienza degli Uffici. Il Senato è una macchina complessa che si fonda su un dato importante: il patrimonio di dipendenti che in essa sono presenti e vi lavorano. Ritengo fondamentale investire in futuro maggiori risorse per favorire e potenziare la strumentazione a disposizione, per la qualificazione, l'arricchimento e l'aggiornamento professionale di coloro che operano all'interno di questa Istituzione. Avere, infatti, dei servizi importanti e qualificati per un parlamentare che si accinge a esaminare un provvedimento legislativo è indispensabile e, pertanto, chi fornisce questi strumenti deve essere sempre al meglio delle proprie possibilità. Dunque, sono indispensabili competenza, aggiornamento, serietà professionale e analisi dei fabbisogni organici. Occorre poi programmare, laddove necessario, l'incremento del personale in organico, prevedendo concorsi unici con la Camera per il reclutamento di nuovo personale. Penso che si debba lavorare, inoltre, per rafforzare ulteriormente i meccanismi di trasparenza dell'Istituzione. In tale ambito, il Gruppo Partito Democratico del Senato rivendica un ruolo primario, rispettoso delle determinazioni assunte negli scorsi anni dal Senato, in termini di trasparenza e pubblicità del proprio bilancio, sempre certificato da revisori esterni. Sempre in tema di trasparenza, occorre lavorare per far sì che il bilancio interno del Senato sia corredato in futuro da un sempre più elevato numero di informazioni, che illustrino nel dettaglio le singole voci di entrata e di spesa. Ciò, al fine di rendere il Senato una casa di vetro, accessibile a tutti i cittadini, anche nelle pieghe più nascoste. Mi avvio alle conclusioni. Quelli delineati sono soltanto alcuni dei possibili interventi per migliorare ulteriormente il funzionamento del Senato e, più in generale, delle istituzioni parlamentari. È un campo d'azione oltremodo necessario, tenuto conto dei numerosi sforzi e sacrifici che tutta la collettività nazionale è stata chiamata a mettere in atto in questi ultimi anni. un ringraziamento particolarmente sentito al Segretario Generale, dottoressa Serafin, ai Vice Segretari Generali e ai Direttori dei Servizi. Si tratta di un ringraziamento che vuole significare l'apprezzamento per il lavoro compiuto, oltre che un attestato di profonda fiducia. Al Collegio dei Questori, anche sulla spinta delle determinazioni che assumerà l'Assemblea del Senato, spetterà formulare nei prossimi mesi le proposte che illustrino il percorso e le iniziative per proseguire nella complessiva riorganizzazione delle nostre istituzioni istituzioni parlamentari. Credo che queste sottolineature dovessero essere fatte con orgoglio e per questo motivo il Gruppo Partito Democratico voterà a favore favore del rendiconto 2017 e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2018. In conclusione, voglio rimarcare un fatto che rimane per noi una ferita aperta:

un elemento positivo, e nella direzione non del controllo, ma soprattutto della garanzia. Le opposizioni devono essere tenute in considerazione e crediamo che questo sia un fatto importante. La ferita è ancora aperta.

secondo noi - sono state calpestate delle prerogative dell'opposizione che, nella gestione

Mi riferisco, in particolare, a dati molto significativi che riguardano la trasmissione telematica degli atti parlamentari mediante la firma digitale, che ha comportato una riduzione considerevole dell'utilizzo della carta, con un risparmio di quasi 5 milioni di euro, grazie al processo di dematerializzazione, sicuramente necessario e doveroso. Visto che da legislatori lo stiamo

modo, apprezziamo le scelte su nuovi investimenti che riguardano, in particolare, la riqualificazione e l'efficientamento energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche il potenziamento della ricerca della documentazione e dell'aggiornamento professionale del personale. Questo significa che, accanto a una riduzione della spesa, c'è comunque una capacità di Questo può sembrare un atto formale, ma credo che non lo sia.

È ovvio che dobbiamo prestare analoga attenzione nel gestire le risorse che vengono affidate al funzionamento del Senato della Repubblica. vengono a volte definite costi della politica, mentre noi riteniamo si tratti - invece - dei costi del funzionamento della democrazia. Se però vogliamo far passare questo messaggio e non far prevalere la demagogia, dobbiamo prima di tutto essere chiaramente responsabili di come gestiamo questi fondi. Noi quindi ci auguriamo che anche nei prossimi anni, i bilanci di previsione approvati dal Collegio dei Questori e dal Consiglio di Presidenza, si continui sulla strada tracciata. È ovvio che risparmiare su grandi cifre stanziate - come avvenuto otto anni fa - e invertire il percorso è più facile, perché tagliare all'inizio comporta la possibilità di incidere effettivamente su spese superflue, che potevano essere contenute e dovevano essere ridotte.

di continuare su questa strada, ovviamente con le dovute attenzioni. Non deve esserci una riduzione della qualità del servizio garantito, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività legislativa.

attenzione e responsabilità. Non dobbiamo deludere le aspettative dei cittadini e dobbiamo continuare su questo percorso, e siamo certi

Signor Presidente - come ha sottolineato più volte - il Senato è al servizio dei cittadini e deve innanzitutto svolgere nel modo migliore il suo compito, che è quello di rappresentare i cittadini, di legiferare di svolgere un'azione di controllo sul Governo e sulle istituzioni in generale, essendo composto, per l'appunto, da rappresentanti eletti direttamente dal popolo. Per fare questo, è indispensabile

studio per rendere il Senato più efficiente nel servire in modo preciso e doveroso il Paese. L'azione svolta dai Questori nei primi mesi della legislatura è andata sicuramente in questo senso.

ancor più, della voce relativa ai senatori (sia quelli in carica, sia quelli non più in carica), abbiamo una tendenza della spesa che, se fosse stata la stessa da parte dello Stato in generale, oggi, anziché parlare di *deficit* più alto o più basso, dovremmo discutere di come impiegare i molti miliardi di avanzo che avrebbero le casse dell'Amministrazione dello Stato.

Per raggiungere siffati risultati, che godono dell'appoggio di tutti, nel corso degli anni sono state tante le mozioni, i suggerimenti e le proposte avanzate per andare in tale direzione.

È doveroso ricordare il lavoro che quotidianamente viene svolto dalla struttura del Senato, dal segretario generale, dottoressa Serafin, ai vice segretari generali presenti, Toniato e Sandomenico, e a tutta la struttura del Senato. *(Applausi dai Gruppi a quest'opera che viene prestata senza badare a orari e senza limiti, sempre al servizio delle decisioni politiche e della conduzione politica data a questa Assemblea. È un aspetto estremamente importante importante e fondamentale, come ha già sottolineato il presidente Schifani, che ha parlato prima di me. Sappiamo che la struttura del Senato è di tale qualità che spesso

essere complesso, ma fatto con grande impegno.

colleghe e colleghi, non ritornerò neppure io sui dati aridi del bilancio interno. In un momento di riduzione complessiva della spesa, è necessario sottolineare alcuni aspetti come l'aumento degli stanziamenti per l'attività di studi e ricerche; il rafforzamento alle attività interparlamentari

Grazie,

all'adeguamento degli edifici del Senato in senso più moderno e innovativo, con un occhio al risparmio energetico, all'ambiente e al superamento delle barriere architettoniche (una fattispecie fondamentale per un edificio pubblico e tanto più per la Camera alta di questo Paese).

Peraltro, mentre credo sia sostanzialmente prevedibile che figure apicali di un'Amministrazione importante, forse una delle più importanti del Paese, abbiano competenza, capacità, oltre che abnegazione al lavoro, non è così facile e scontato trovare il senso

a conclusione dell'esame dei documenti finanziari e prima della votazione finale, vorrei anch'io intervenire per esprimere un ringraziamento sentito ai senatori Questori per l'impegno solerte e proficuo nel cercare di soddisfare al meglio le numerose e articolate esigenze di funzionamento di questa Istituzione. Con questo progetto di bilancio il Senato ha inteso dare un chiaro segnale nella direzione di una spesa sempre più razionale e ispirata ai principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità. Ai senatori Questori va dunque riconosciuto il merito di aver saputo perseguire una virtuosa opera di contenimento dei costi, senza tuttavia rinunciare all'opportunità di implementare gli investimenti in settori strategici, con interventi sia relativi alla sostenibilità energetica e funzionale degli edifici del Senato, sia mirati a una costante crescita delle professionalità e delle attività di studio e di ricerca. Ringrazio inoltre il Segretario Generale, l'Amministrazione che rappresenta e il personale tutto, che hanno quotidianamente reso possibile il conseguimento degli ambiziosi obiettivi che si sono prefissati. *(Applausi)*. Grazie, grazie davvero.

Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente. Nella seduta di domani e nella seduta di giovedì 6, che non prevede orario di chiusura, saranno discussi la mozione sulla tutela del settore agroalimentare italiano, la legge europea 2018 e il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio in materia di concretezza delle pubbliche amministrazioni. Resta altresì confermato per giovedì 6 alle ore 15 il *question time*, con i ministri Centinaio, Toninelli e Costa. Lunedì 10 dicembre, alle ore 17, il Presidente renderà le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto della legge di bilancio. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro le ore 19 di mercoledì 12 dicembre. L'Assemblea si riunirà inoltre mercoledì 12 dicembre, alle ore 15,30, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei dei ministri in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018. L'ordine del giorno della seduta, senza orario di chiusura, potrà inoltre prevedere l'eventuale Grazie a tutti della settimana prevede seduta anche venerdì 14 dicembre, se necessario. Nella settimana successiva, con sedute senza orario di chiusura a partire da martedì 18 fino a sabato 22 dicembre, se necessario, sarà discusso il disegno di legge di bilancio.

alla Conferenza dell'ONU sull'emigrazione a Marrakech. Per la verità, vorrei ricordare in

dell'accordo o comunque aveva annunciato che avrebbe sottoscritto il documento e che avrebbe partecipato alla Conferenza di Marrakech. Cosa sia cambiato da due mesi a questa parte non è dato saperlo, però il presidente del

ritiene opportuno parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte all'esito di tale discussione, però l'Italia non parteciperà alla Conferenza. Alla luce di questa breve premessa, noi abbiamo chiesto, insieme anche ad altri Gruppi, di avere la possibilità di parlamentarizzare il dibattito, cioè di avere la discussione in Parlamento, in particolare nell'Aula del Senato, con comunicazioni o del Presidente del Consiglio o del Ministro degli esteri, e una una presa di posizione attraverso la votazione di risoluzioni in vista della Conferenza di Marrakech. Per la verità, per come sono organizzati i nostri lavori, credo che noi avremmo tranquillamente la possibilità di approfondire. Infatti, questa settimana si può approfondire nella Commissione esteri e, contemporaneamente, possiamo calendarizzare - questa è la proposta secca che faccio - le comunicazioni,

sui cambiamenti climatici. I dati, rilanciati anche da questa Conferenza e poche settimane precedenti anche dall'ultimo rapporto IPCC dell'ONU, sono molto

a Parigi e se confermeremo l'impegno per il raggiungimento della neutralità energetica nel 2050 annunciato dall'Europa, siccome ci mancano una serie di elementi (non sappiamo, ad esempio, che fine abbia fatto il piano di adattamento ai cambiamenti climatici), avevamo chiesto un'informativa, ma anche su questo si è rinviato tutto al mese di gennaio, sperando che, nel frattempo, non si verifichino altri disastri

Conferenza dei Capigruppo, terminata prima dell'inizio dei lavori di quest'Aula, abbiamo avanzato una proposta di calendario diverso da quello poi assunto dalla Conferenza. Intervengo, dunque, per ribadire le nostre posizioni e per integrare il calendario con le proposte che avevamo già avanzato.

Ovviamente, ci siamo accorti tutti che proprio la prossima settimana, nelle giornate del 10 e dell'11 dicembre, a Marrakech si terrà una importante Conferenza sul tema, quindi chiediamo coerenza e rispetto per queste istituzioni e chiediamo che il Governo,

luce di ambigue affermazioni che vengono riportate dai *media* in questi giorni, affermazioni del Governo. La motivazione del mio intervento, ovvero la proposta politica riguarda il fatto che abbiamo chiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo, tramite il presidente Marcucci - e lo chiediamo ancora oggi - che il ministro Di Maio venga in Aula per informare il Parlamento sulla triste vicenda che da giorni è ripresa, ahimè, da tutti i *media* nazionali, che riguarda la sua famiglia, la sua azienda

io ho voluto essere essenziale ma non certo per alleggerire la gravità di questa vicenda. Mai, io credo e noi riteniamo, che il Parlamento si possa e debba sostituire alle prerogative dell'autorità giudiziaria, ma nemmeno può abdicare al suo ruolo di responsabilità politica e di vigilanza sull'attività del Governo. Non esiste una ragione per cui quest'Aula non chieda al ministro e vice presidente Di Maio di venire in Senato a chiarire la sua posizione personale relativamente alle vicende di cui sopra. confidiamo di avere celermente una risposta su questo punto e che il Ministro possa venire in Aula già nei prossimi giorni. Rispetto invece alla proposta di integrazione del calendario e di modifica,

quindi invitando il Governo a non ratificare questa intesa, perché noi abbiamo preso sul serio la valutazione del Governo di parlamentarizzare, com'è assolutamente corretto, la discussione Francamente riteniamo che i tempi ci siano, sia nel corso delle sedute di questa settimana, anche oggi stesso, dato che la seduta sta per terminare

anche lunedì. La nostra richiesta è rilevante proprio perché il vice presidente del Consiglio, senatore Salvini, alla Camera - perché non ho ascoltato Grazie,

condizione specifica dell'Italia, quale Paese proteso nel Mediterraneo, con i problemi migratori che conosciamo e non devo qui richiamare, abbia interesse a valutare in anticipo cosa fare. L'agnosticismo, cioè dire «Non vado», come dice Conte, «perché non mi ci mandano», sostanzialmente, o «perché non so che dire», non è una posizione seria. È noto che io non la penso come la senatrice De Petris, che pure chiede, con motivazioni diverse dalle mie, la discussione di questo tema, ma il Parlamento e la democrazia servono a questo: le decisioni si prendono nelle Aule parlamentari, non al telegiornale!

ma una discussione a babbo morto o a Marrakech celebrato ha poco senso e non è decoroso avere un Presidente del Consiglio che si rimangia quello che ha detto e non va. Abbia il coraggio di affrontare l'Assemblea e dire quello che pensa. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Noi non vogliamo firmare quella convenzione, ma vogliamo che il Parlamento sovrano

ma in un momento di democrazia parlamentare potrebbero emergere posizioni di maggiore omogeneità. Insistiamo convintamente e lo diremo dentro e fuori il Parlamento, perché non è che si fanno gli annunci alla Camera e si impedisce alle Camere di votare sul tema.

Se non fosse stato per le battaglie di Fratelli d'Italia, di tutto questo non si sarebbe saputo nulla: il Global compact sarebbe stato firmato il 10 dicembre a Marrakech nel totale silenzio dei grandi media, delle istituzioni e del Parlamento tutto, perché nessuno aveva speso una sola parola su di esso*.* È stato Fratelli d'Italia a imporre a tutto il Paese la discussione sul tema e ne siamo fieri. Siamo contenti che finalmente la questione sia diventata di

l'impostazione delle Nazioni Unite e, di conseguenza, dei singoli Stati, da qui al futuro, in tema di immigrazione. Il Global compact for migration è un documento pericoloso, perché inserisce una serie di ovvietà, la tutela dei diritti umani e del migrante, già ampiamente presenti in tutte le convenzioni internazionali in tema di migrazione e in tema di diritti umani. In tutto questo inserisce però delle novità la novità è, di fatto, il diritto fondamentale a migrare e l'obbligo, di conseguenza, degli Stati di non limitare questo diritto fondamentale dell'essere umano. Con il Global compact for migration si sancisce la fine delle frontiere e degli Stati nazionali, l'immigrazione incontrollata e illimitata: questo è il Global compact ed è per questo che una serie di Stati, come gli Stati Uniti, l'Austria, l'Australia, Israele, la Slovacchia, la Svizzera e ogni giorno se ne sommano di più, non parteciperanno alla convenzione di Marrakech e non firmeranno il Global compact L'Italia fino a ieri aveva dichiarato che avrebbe firmato il Global compact: lo ha detto il Presidente del Consiglio. Anche su questo noi ci dobbiamo capire: chi è il Presidente del Consiglio? Il problema è che questo tema non è secondario. Fratelli d'Italia ha chiesto, alla Camera, di discutere il Global compact for migration prima del 10 dicembre e ci è stato risposto che verrà calendarizzato la notte di Natale: il 23 dicembre si discuterà del Global compact: una cosa assolutamente ignobile! Al Senato abbiamo formalizzato in ogni sede la proposta di discutere di questo prima del 10 dicembre, del 10 dicembre, ma ci è stato risposto di no, poche ore fa, alla Capigruppo, non è stata accettata la nostra mozione e si parlerà di tale questione dopo la Conferenza di Marrakech del 10 dicembre. chiede che la discussione sia fatta prima del 10 dicembre, perché questa Assemblea e il Governo su questo tema non possono continuare a fare il gioco delle tre carte: devono dire se sono a favore dell'invasione delle nostre frontiere o se sono contrari. Continuare a fare melina su questo, non pronunciarsi e continuare ad avere il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri che dicono di essere favorevoli a questo trattato,

è paradossale che, pur pensandola sul Global compact for migration in modo completamente opposto ai colleghi di Fratelli d'Italia, devo dire che hanno ragione. Qui c'è un problema che riguarda il rapporto tra il Parlamento e il Governo. Noi siamo una Repubblica parlamentare, il Governo parla con lingua biforcuta su un problema fondamentale e noi siamo espropriati della possibilità di decidere nei tempi desiderati e giusti. Abbiamo una presa di posizione del Ministro degli esteri, che si è dichiarato disponibile a venire in Parlamento, allora, colleghi, voglio capire: se sono cose formali e sulla politica estera si viene a riferire in Parlamento solo sulle cose ovvie, magari per leggere quello che noi sappiamo benissimo perché l'abbiamo letto sui giornali, giornali, queste informative non servono assolutamente a nulla. Se c'è un punto su cui il Parlamento non può essere espropriato del diritto-dovere di decidere, questo è il Global compact, che credo - consentitemi di dire solo questo in pochi secondi - che molti dei nostri colleghi non abbiano letto, perché se pensiamo che tale accordo sia una minaccia per la sovranità nazionale,

oggi: sarà la sede adatta il giorno in cui sarà calendarizzato. Mi associo a quanto ha detto il Gruppo del PD nella persona del senatore Ferrari: o come informativa urgente o come comunicazione del Governo, credo sia fondamentale che il Parlamento si riappropri del suo diritto-dovere di decidere. Aggiungo anche che nella storia della Repubblica siamo pieni di posizioni che vedono una divaricazione all'interno del Governo, che due *partner* del Governo la pensano diversamente. Se facessimo finta di indignarci perché la Lega e i 5 Stelle la pensano diversamente, vorrebbe dire che non abbiamo assistito negli ultimi trent'anni a quello che è capitato, perché molte volte capita che ci siano posizioni diverse nell'ambito dello stesso Governo. Tuttavia qui il dato è diverso: loro comporranno come ritengono la loro maggioranza, ma noi non possiamo essere espropriati del diritto di decidere e questo non può avvenire quando i giochi sono già fatti e il nostro Governo si è associato alla Svizzera (aperta parentesi, punto esclamativo, puntini puntini, chiusa parentesi). Io credo che noi dovremmo, oggi, con questo voto sul calendario, riappropriarci del nostro diritto-dovere.

entro il 10 dicembre, ma non perché si voglia impedire o espropriare il Parlamento di un suo diritto, bensì perché riteniamo che, alla luce delle dichiarazioni fatte dal Governo, che ha detto che non parteciperà di Marrakech, non si capisce per quale motivo dovremmo venire qua ad esprimerci per indirizzare il Governo sul vertice di Marrakech. Se non partecipa, non c'è bisogno di indirizzarlo e quindi non c'è tutta questa fretta e questa urgenza di dover calendarizzare

però, se vogliamo approfondire il tema, dato che ho sentito dire che bisogna studiare prima di capire cosa dice il Global compact, studiamo e approfondiamo: vogliamo limitare un tema così importante, un trattato internazionale,

pertinente e competente per materia. E vogliamo dimenticarci la Commissione affari esteri? Certo che no, anche lì bisognerà fare le congiunte! Ma visto che si parla di migrazione, forse ci sono anche altre Commissioni che possono essere coinvolte. Ecco, questo è il modo

c'è la manovra economica, c'è il disegno di legge anticorruzione, abbiamo un calendario fittissimo e ne abbiamo preso atto tutti,

invece dovremmo ringraziare il Governo per aver deciso di parlamentarizzare le decisioni che saranno prese su un trattato così importante come il Global compact infatti che ci sia una dignità di quest'Assemblea che vada rispettata e anche che vada rispettata quella della Camera dei deputati. È una discussione che dovrà camminare di pari passo ed è una decisione che verrà presa dal Parlamento nella libertà della scelta che poi ciascun Gruppo parlamentare farà e mi rivolgo, per il tramite della Presidenza, al collega Casini, che potrà partecipare a quel dibattito e prendere le decisioni che riterrà opportune. Poi, se saranno quelle della maggioranza, avranno ovviamente il favore del voto, se saranno invece quelle minoritarie nelle Aule parlamentari, verranno ovviamente respinte. Non vedo dove sia il problema nel dire che spostiamo questa discussione importante in un momento in cui si possa affrontare con l'importanza che merita

la provocazione - la chiamo così - del Partito Democratico di chiedere al ministro Di Maio di venire in Aula a riferire di un tema che, con la sua attività di parlamentare e con la sua attività di Ministro, non c'entra nulla ed è un problema che è già stato ben chiarito in tutte le sedi opportune,

Non si è mai nascosto e, anzi, ha cercato di accompagnare e agevolare quelle indagini e quei momenti di giornalismo d'inchiesta che forse troppo spesso sono mancati in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi M5S e* *L-SP-PSd'Az)*. Quindi ritengo che abbia fatto molto bene a chiarire, dove doveva chiarire, ma non è certo questa la sede dove deve farlo.

che i Ministri si sono espressi pubblicamente sulle questioni che sono state qui sollecitate, ma la funzione del Parlamento è, per l'appunto, quella di essere l'organismo davanti al quale i Ministri rendono conto con contraddittorio, con la possibilità del Parlamento di esprimersi. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

il senatore Gasparri, o attraverso l'esame delle mozioni o a seguito delle comunicazioni del Ministro competente.

Grazie,

per rappresentare, ancora una volta, il problema delle mafie che operano in provincia di Foggia. Oggi intervengo per dare buone notizie, ma purtroppo anche due notizie meno buone, anzi decisamente cattive.

l'auto del comandante della stazione dei Carabinieri di Cerignola, il capitano Michele Massaro. Ovviamente a loro va la mia e la nostra solidarietà; ho espresso analoga solidarietà

voglio essere più preciso: venerdì 30 novembre sono stati eseguiti 30 arresti a Foggia di presunti appartenenti ai clan mafiosi. È la più grande operazione che abbia riguardato clan di mafia Grazie a tutti appartenenti a un clan mafioso, ritenuti della mafia garganica; mercoledì 28 novembre, invece, erano stati eseguiti 14 arresti a San Severo. Siamo ovviamente molto soddisfatti che si sia imboccata questa strada e esprimiamo il nostro plauso e il nostro sostegno pieno agli investigatori, alle Forze dell'ordine e ai magistrati. *(Applausi

Signor Presidente, una recente sentenza del Consiglio di Stato ha dato ragione a Enel e torto al Forum ambientalista nazionale e a ISDE-Italia, Medici per l'ambiente, circa la mega centrale Enel della Valle del Mercure, situata nel cuore del Parco nazionale del Pollino, tra Calabria e Basilicata. Si tratta di un impianto che brucia 350.000 tonnellate di alberi ogni anno, trasportati da oltre 100 TIR al giorno. Di fatto, la sentenza si basa su un parere del Consiglio dei ministri presieduto da Matteo Renzi, a cui la Regione Calabria, governata da Mario Oliverio, ha chiesto di intervenire per superare il parere ostativo del direttore dell'ente Parco del Pollino. Matteo Renzi ha risposto «presente», non dando alcun peso al fatto che la centrale non ha l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ha la valutazione di incidenza (VI) scaduta e che Enel, nel progetto, ha addirittura presentato dati di una valle diversa da quella del Mercure. Senza dimenticare che parliamo di un'area ultraprotetta, essendo parco nazionale, zona di protezione speciale dell'Unione europea e patrimonio dell'umanità UNESCO. Neanche Matteo Renzi ha avuto il coraggio di prendersi tutta intera questa responsabilità, cosicché il Consiglio dei ministri ha dato parere positivo, subordinandolo però a una deroga del Piano del parco in via di approvazione, che boccia, in uno specifico paragrafo, proprio la centrale del Mercure. La Regione Calabria del presidente Oliverio, forte di questo parere, ha dato comunque l'autorizzazione, senza attendere alcuna deroga. La lotta del forum Stefano Gioia (che, a fianco delle popolazioni della Valle del Mercure, sedici anni combatte contro questa aggressione al territorio, alla salute e all'occupazione vera, legata al turismo e all'agroalimentare di qualità) continua senza sosta, anche in opposizione alla 'ndrangheta, che ha infiltrato la fornitura di biomasse alla centrale.

Il MoVimento 5 Stelle, che è stato per anni in prima linea contro la centrale del Mercure, ha - io credo - l'obbligo di dare concretezza al suo impegno e ai suoi impegni, stroncando, finalmente, uno scandalo creato e gestito dalla vecchia politica sulla pelle dei cittadini e a danno di un territorio protetto

Il ministro Grillo ha revocato la nomina dei componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità, l'organo tecnico-consultivo più importante del Ministero della salute. Si apprende con stupore la decisione di tali revoche, posto che, come dichiarato da quasi tutti i membri revocati e come risulta, il ministro Grillo non ha mai incontrato il Consiglio superiore della sanità, né ha mai richiesto alcun parere, né altra attività di supporto. La notizia ha scosso tutto il mondo scientifico e della sanità, apparendo la decisione assolutamente arbitraria e priva di alcun fondamento. Se è vero, infatti, che trattandosi di un organo consultivo e di supporto che coadiuva il Ministero della salute, è pur vero che - giuridicamente e politicamente - la discrezionalità non coincide con l'arbitrio e l'uso arbitrario e ingiustificato del potere. È diritto di tutti i cittadini, per il tramite di noi parlamentari, conoscere le ragioni e le motivazioni di simili brutali scelte, che potrebbero apparire come dettate da logiche perverse di parte in una materia come la salute pubblica, che ha bisogno, invece, di oggettività e scientificità per la superiore tutela dei pazienti. Presidente, chiediamo che il ministro Grillo venga in Aula per esporre quali siano le motivazioni gravi delle revoche, come intenda sostituire i membri revocati e se tale scelta non sottenda un esercizio di potere finalizzato limitatamente alle battaglie del suo partito di appartenenza e non all'interesse comune del nostro Paese e del diritto alla salute dei nostri cittadini, che

di minoranza sul disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" concernente la "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018" e la "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017"